che a 20 chilometri dal centro del cratere ci sia stata una casa che ha subito forti anni. Bisogna però fissare le priorità, signor Sottosegretario,

spesso in nome dell'emergenza si fanno le più grandi storture nella gestione. Credo che invece dovrebbe essere sancita per legge che vi sia un'intesa istituzionale quando si tratta di programmazione. Il commissario delegato è chiamato a mettere in atto azioni amministrative celeri, ma non può, nella maniera più assoluta, superare superare il compito primario di un pubblico amministratore, cioè quello di programmare sul proprio territorio: bisogna essere celeri, ma non si deve assolutamente scippare la programmazione agli eletti

poi all'emendamento 1.313, ho notato che durante la gestione del terremoto manca la fase di controllo,

è quello di non creare situazioni italiche dove questi allargamenti sono stati realizzati a dismisura. Il problema riguarda tutti quei soggetti che abbiano effettivamente subito danni, diretti o indiretti, in conseguenza del sisma, quindi collegati con un nesso di causalità con l'evento sismico del 6 aprile. Nell'attuale formulazione, signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, i Comuni nel cui territorio si fossero realizzati danni in conseguenza del sisma

con un provvedimento amministrativo *ex* comma 1 dell'articolo 1, il commissario delegato o il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, inserissero

cui ogni soggetto ed ogni comunità che abbiano subito un danno, diretto o indiretto, in conseguenza del sisma, abbiano diritto al risarcimento. la verifica del danno e l'entità del risarcimento o della modalità del contributo possono dipendere unicamente dall'ordinanza, cioè dal provvedimento amministrativo del sottosegretario Bertolaso, in quanto commissario delegato,

attuale, fuori dall'elenco dei Comuni del cratere non ha diritto a nulla. Se il Sottosegretario e il relatore accedessero ad un'interpretazione corretta

illustro l'emendamento 1.308 perché, per le ragioni che sono state espresse anche dai colleghi che mi hanno preceduto, i senatori Astore e Lusi, per noi dell'Italia dei Valori è fondamentale per definire una certezza di diritti per tutte le popolazioni e le comunità che sono state colpite dal terremoto.

in questo Parlamento, di correggere quelle storture e quelle mancanze che non avrebbero alcuna giustificazione. Ricordo c'è una contraddizione di fondo tra la disposizione di legge che riserva la delimitazione del cratere sismico ai Comuni colpiti dal sisma pari o superiore al sesto grado della scala Mercalli e quando si dice che

è un invito al ritiro poiché la materia della comunicazione al Parlamento su tutte le iniziative intraprese dal commissario delegato dal Governo è affrontata in altra sede ed e già stato approvato in Commissione un emendamento che prevede la cadenza semestrale delle informative. Esprimo parere contrario sull'emendamento

il suo emendamento si riferiva al comma 1 dell'articolo 3. Comunque, in presenza della riformulazione dell'articolo 3 proposta dalla Commissione - che mantiene peraltro il richiamo dello stesso articolo 3

della normativa antisismica, più volte proposta dal Governo e approvata dal Parlamento, se attuata nei termini approvati dalla Commissione travolgerebbe pure tutte le precedenti revoche; è quindi più corretto dire che c'è un nuovo termine, che poi è quello prossimo del 30 giugno e corrisponde sicuramente alla volontà espressa da tutte le componenti parlamentari presenti in quest'Aula,

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.301 sulla rendicontazione della gestione commissariale, vi sono già

A proposito dell'emendamento 1.600 e relativi subemendamenti chiederei un accantonamento, perché è *in itinere* una riformulazione da parte del Governo

la Protezione civile. Credo che sia stato svolto un buon lavoro; mi sono recato spesso a Napoli nell'ultimo periodo e ho trovato una situazione ordinata sotto il profilo della raccolta dei rifiuti.

Mi sembrava assolutamente naturale che il Governo e il relatore accedessero alla richiesta che i provvedimenti del commissario vengano motivati, che siano trasparenti e sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Emendamenti studiati e mirati perché non interferiscano in alcun modo con le attività di soccorso della Protezione civile, in occasione del terremoto che ha

contrario del relatore e del Governo mi fa pensare che esistano delle ragioni di fondo, delle motivazioni politiche per le quali questi emendamenti non vengono accolti.

il sottosegretario Bertolaso riveste contemporaneamente la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e la carica di Capo del Dipartimento della protezione civile. Credo che questo sia un errore che indebolisce fortemente il credito di cui il sottosegretario Bertolaso ha bisogno per svolgere la sua missione. Oggi il Sottosegretario non è in Aula, signor Presidente, perché giustamente sta lavorando in Abruzzo per cercare di risolvere i gravissimi problemi causati dal terremoto. È giusto che sia in Abruzzo come Capo della Protezione civile, ma come Sottosegretario dovrebbe stare invece in Aula, perché compito del sottosegretario è essere presente in questa sede

capo dipartimento o direttore generale di un Ministero. I motivi di fondo riguardano la distinzione tra la pubblica amministrazione e l'attività del Governo. La pubblica amministrazione, per dovere costituzionale, è tenuta all'imparzialità; il Governo, per la sua natura, è tenuto ad esprimere un indirizzo politico. Invito quindi il presidente Berlusconi e il sottosegretario Bertolaso, nei confronti del quale ho molto rispetto e anche apprezzamento per il suo lavoro, a riflettere su un cumulo di cariche

chiedesse di fare il Sottosegretario all'interno, se il Segretario generale del Ministero degli affari esteri chiedesse di fare il Sottosegretario agli esteri o se il capo di stato maggiore chiedesse di fare il Sottosegretario alla difesa. Sono anomalie, signor Presidente, che vanno sanate. Come credo che vada sanata un'altra anomalia e cioè l'eccesso delle competenze della Protezione Abbiamo bisogno di una Protezione civile che si occupi di protezione civile e di emergenze; non vedo per quale motivo debba occuparsi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dell'incontro internazionale per la pace a Napoli, dell'Expo di Milano, della visita del Papa ad Assisi e potrei continuare. Credo, signor Presidente,

Il sottosegretario Bertolaso, di cui ho grande considerazione, si è occupato della preparazione del Giubileo (e, ne ho avuto personale conoscenza, lo ha fatto in modo egregio), evento di gran lunga superiore, per impegno, dimensione e complessità, a tutti gli altri eventi che prima ho citato ed agli altri che potrei ancora citare. Credo, signor Presidente, che il Giubileo del 2000 sia stato ben organizzato a legislazione ordinaria, senza modifica alcuna alle leggi dello Stato e che questo si possa fare anche per gli eventi che ho appena nominato. Vorrei aggiungere un'altra questione. Ho chiesto agli uffici del mio Gruppo di farmi conoscere quali sono le norme di legge che possono essere che possono essere ignorate dalle ordinanze della Protezione civile. Non sono in condizioni adesso di leggere

di una pagina di articoli del codice degli appalti, di mezze pagine di norme sul procedimento amministrativo, sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato,

a parte i possibili problemi di costituzionalità (mi chiedo infatti come nel nostro ordinamento possa esistere una legge che autorizza atti amministrativi successivi ad aggirare un pacchetto così consistente di norme

diversa tipologia di ordinanze nel nostro ordinamento. Quello che dice il senatore Zanda è nella legge autorizzativa delle ordinanze; se noi dicessimo oggi che queste ordinanze hanno bisogno di tali accorgimenti, di tali accorgimenti, implicitamente autorizzeremmo la possibile emanazione di ordinanze che non ne hanno. Queste sono le caratteristiche delle ordinanze previste dalla Protezione civile in regime di emergenza.

della Corte dei conti e di tutti gli organi istituzionalmente preposti ai controlli. Diversamente, ripeto, potremmo rischiare di fissare due livelli di ordinanza, il che, a mio avviso, non è opportuno.

relativamente alla disposizione del comma 3 dell'articolo 1, che definisce, per così dire, lo *status* dei Comuni terremotati, ma fuori dal cratere sismico così come individuato con ordinanza della

il Governo ha presentato un emendamento in cui il contributo per la ricostruzione delle abitazioni è totale senza modificare di una virgola la copertura. Ecco perché forse è bene parlare chiaro: vogliamo continuare a mantenere un atteggiamento di collaborazione e di proposta, soprattutto chi ha vissuto in prima persona un altro terremoto, ma non vogliamo nella maniera più assoluta essere emarginati e tacciati di non fare gli interessi delle popolazioni abruzzesi.

due semplici ragioni, di cui la prima è di natura tecnica. Oggi il Governo presenta il nuovo aggiornamento al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro; lavoro; questo emendamento, che è a costo zero, non fa altro che ribadire la necessità che, nonostante l'accelerazione dei tempi, nonostante la situazione emergenziale, e al di là della possibilità

sta avvenendo un ampio dibattito sulle necessità, sulle misure e sui controlli da apportare. La fase del post-terremoto potrà determinare infatti elementi di grave stortura, con infiltrazioni anche di delinquenza organizzata che potrebbero avvelenare il clima della ricostruzione. Il Parlamento oggi è pertanto chiamato semplicemente ad introdurre un elemento che noi consideriamo lapalissiano nella costruzione di questo provvedimento legislativo. In secondo luogo, la ragione politica per la quale non si può ritirare un emendamento è altrettanto evidente: se si rifiuta

questo precluderebbe ogni possibilità da parte delle opposizioni di introdurre qualsiasi altro elemento migliorativo e correttivo allo stesso disegno di legge; quindi il nostro lavoro

nella fase del post-terremoto ad un grande senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, e chiedo che l'emendamento sia messo ai voti

è ineludibile la necessità di fare delle scelte rapide ed immediate, dal momento invece di attuazione anche della della prima fase di ricostruzione, quella che è stata chiamata «la ricostruzione leggera». Prevediamo dunque che la Conferenza dei servizi proceda in accordo e in coordinamento con le amministrazioni provinciali e comunali

Sappiamo bene che è probabile che, per accelerare sui tempi, si debba far ricorso ai *general contractor*, i quali poi, a loro volta, procederanno ad un subappalto in deroga, nei termini del 50

e sottovalutarla è da irresponsabili. Sto sottolineando questo aspetto perché per la prima volta oggi su un giornale -non mi era finora mai accaduto - leggo le considerazioni di un tecnico stimato

che sul tema della *governance* c'è un'esigenza pressante, come lo stesso presidente Marini riconosceva, e anche un'assunzione di responsabilità forte da parte del Governo per le fasi dell'emergenza, che non è terminata e che terminerà quando avremo messo

notevoli passi avanti verso un'intesa sulla *governance* e noi stessi riconosciamo l'assoluta legittimità degli enti locali a riprogrammare il loro territorio. Credo che il Governo stia per presentare un emendamento aggiuntivo al comma 13 dell'articolo 2 - di questo pregherei, non appena arrivato, di darne notizia anche ai colleghi, oltre che al relatore

esclusivamente per i centri storici, ma per l'intero territorio comunale. Quindi, pur comprendendo le argomentazioni del presidente Marini, credo che lo stesso, così come gli altri colleghi, debbano comprendere anche le argomentazioni di

al commissario delegato e quindi al Governo, che se ne assume l'intera responsabilità. L'impostazione del Governo è pertanto quella da mantenere e quindi la più corretta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

«I Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il Presidente della Provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo una armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1».

molto delicato delle indennità di espropriazione delle aree occupate per la realizzazione di moduli abitativi e di quelle che necessiteranno per sopperire alle altre esigenze. Poiché su questo tema, proprio in questi giorni e in queste ore vi è una vera e propria sollevazione, come alcuni colleghi sanno, da parte dei proprietari espropriati, vorrei chiarire qual è il punto fatto oggetto dell'emendamento 2.270 e il testo che invece è stato

stabilisce soltanto che il commissario delegato provvede a definire l'indennità di espropriazione senza altro aggiungere, quindi con ogni evidenza facendo riferimento alla legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità. La Commissione, su proposta dei colleghi della maggioranza, ha inteso aggiungere (ed è questo l'oggetto dell'emendamento 2.270): «tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009»; ovvero, se le aree, come è per gran parte di questi siti occupati o in via di occupazione, avevano una destinazione agricola e comunque non edificatoria, esse andranno indennizzate a valore agricolo, quindi, per pochi euro al metro quadro. Sennonché, come ci è noto, a queste aree viene impressa, con il provvedimento d'urgenza del commissario delegato, una destinazione edificatoria. Ora, si sta verificando, signor Presidente, e mi rivolgo al rappresentante del Governo, che moltissime famiglie, comunque proprietarie di aree terremotate, che hanno ricevuto danni enormi di vario genere, si vedono espropriare, con forma da esproprio proletario vero e proprio, delle aree che noi indennizziamo a 2, 3 o 4 euro, determinando una vera e propria disperazione di queste famiglie. A volte le sottraiamo per ragioni di pubblica utilità e di urgenza, certamente, ma almeno diamo loro il giusto ristoro! Quel ristoro che è stato sancito con una pronuncia recente della Corte costituzionale, che ha stabilito in via definitiva che l'indennità di espropriazione deve essere calcolata al valore venale. Noi proponiamo con l'emendamento 2.270/300 di indennizzare le aree a valore di mercato, così come vengono definite

colleghi, sono sinceramente stupito di questa obiezione, perché lo scopo dell'emendamento 2.270 è quello di ricondurre alla medesima condizione una procedura espropriativa *sui generis*, nella quale l'atto approvativo del progetto comporta la variante urbanistica, quindi la valorizzazione delle aree, rispetto a quanto ordinariamente avviene nei procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche nei quali, come è stato correttamente ricordato, si fa la stima del valore venale del bene espropriato, non già in funzione del bene e dell'infrastruttura pubbliche che si realizzano, ma in funzione della destinazione d'uso in essere rispetto ai piani regolatori in quel momento. Consentire una valutazione in funzione delle opere che si costruiscono nell'interesse primario della popolazione dell'Abruzzo provocherebbe, rispetto a questi espropri rapportati all'ordinario, un indebito arricchimento che credo debba essere preso in considerazione anche per il fatto che l'approvazione dei progetti non certifica l'immediata

di necessità per la collettività e a questo regime è corretto richiamarsi senza avere corsie diverse o, in maniera ancora più discutibile, una diversità di trattamento rispetto a quanto regolarmente avviene.

Signor Presidente, a me fa specie sentire parlare di indebito arricchimento. Noi stiamo parlando di una situazione estremamente delicata. Ci sono alcune decine di persone che vivono della coltivazione dei loro campi.

corrispondendo l'indennità per la destinazione agricola che hanno quei terreni; di cosa dovranno poi vivere queste persone? Stiamo sommando ai drammi altri futuri drammi, non possiamo non farcene carico. Non possiamo ignorare che non stiamo parlando di speculatori, ma di gente che vive del lavoro unico di un'attività agricola: se togliamo loro quel bene dovranno pur vivere in futuro! Come li assisteremo? Altro che indebito arricchimento! Se poi pensiamo che all'articolo 3 sono previsti incentivi e aiuti qualora vi siano state conseguenze economiche per le attività di impresa provocate dal sisma, come non considerare le conseguenze economiche non provocate dal sisma ma dagli espropri delle uniche attività dei nostri concittadini? Mi rivolgo anche al Presidente della Commissione agricoltura: non possiamo essere indifferenti di fronte a questo tema sommare dramma a dramma. E allora, quanto meno indennizziamo tali attività con il valore che si assegna all'area considerandola a destinazione urbanistica e non quale terreno agricolo. Quantomeno, indennizziamo in questo modo;

colpiti indirettamente dal sisma. Questo non lo possiamo consentire, nel rispetto della dignità umana e delle persone, del sacrificio e del lavoro.

mi unisco al suo grido di dolore a soccorso delle popolazione agricola colpita. Peraltro, voglio ricordare a me stesso, al senatore Li Gotti e a tutti i colleghi, che già la legislazione attuale sugli espropri, come ricordava correttamente il senatore Orsi, prevede, nel caso dei piccoli proprietari, dei piccoli contadini, dei coltivatori diretti, gli agricoltori a titolo principale, i cosiddetti agricoltori professionali, sottolineo: tre volte tanto) dell'indennità di esproprio. Aggiungo anche che negli ultimi anni si assiste, almeno nelle Province più evolute, un sostanziale allineamento tra i valori di esproprio stabiliti a livello provinciale e i valori venali di mercato dei terreni agricoli. Lo dico per esperienza diretta.

ragione in linea assolutamente generale) è già prevista, appunto, una triplicazione dell'indennizzo, quindi nessuno viene messo sulla strada. Facciamo un esempio pratico: il coltivatore diretto che viene espropriato dei suoi tre ettari di orto o dei suoi cinque ettari di pascolo

è un documento che attesta l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento e ciò serve a dare la possibilità alle aziende di lavorare in chiaro, di non subire la concorrenza sleale di coloro che si avvalgono del lavoro in nero e a far sì che in Abruzzo si possa fare una ricostruzione sana, veloce e nella trasparenza.

invece che il pagamento avvenga con bonifici bancari e, quindi, che non ci sia passaggio di denaro se non con una sua tracciabilità.

Presidente, vorrei sollecitare una riflessione sull'articolo 3, perché la Commissione bilancio - il presidente Azzollini ne potrà dare atto - ha accantonato l'esame della copertura finanziaria su due emendamenti molto importanti - uno della Commissione e uno a firma di colleghi del Partito Democratico - che attengono alla verifica dell'integrità della copertura finanziaria per gli interventi di ricostruzione con particolare riferimento

Presidente. A seguito di una nostra precisa richiesta, il Presidente della Commissione bilancio ha disposto l'acquisizione di una relazione tecnica integrativa

Per questa ragione, le chiedo di voler disporre l'accantonamento dell'intero articolo 3, in attesa che la Commissione bilancio faccia il suo lavoro,

L'accantonamento dell'emendamento 3.700 e la relazione tecnica richiesta, che va incontro ad esigenze molto giuste poste all'interno della Commissione, tecnicamente non impedisce

È chiaro che l'accantonamento di quell'emendamento impedirebbe il voto finale sull'articolo, ma non su tutti gli altri emendamenti. Questo esclusivamente sotto il profilo tecnico. Per le altre questioni, la decisione naturalmente non compete a me.

nello spiegare la consistenza del problema che ho sollevato. Stiamo parlando dell'aspetto centrale del provvedimento, cioè se ci sono o no le risorse

una nuova relazione tecnica, non comprendo come si possano vagliare gli emendamenti riferiti all'articolo 3. Tuttavia, poiché il nostro intento non è in alcun modo dilatorio né di altro genere, ma è di altro genere, ma è esclusivamente quello di pervenire ad un esame puntuale e informato del provvedimento,

il mio emendamento, che diventa aggiuntivo ad un emendamento approvato già in Commissione, riduce i *quorum* assembleari per decidere la ricostruzione del fabbricato. Questo, al fine di favorirla. Infatti, in caso contrario, potrebbe anche non essere effettuata per l'opposizione

che già disciplinano queste situazioni potranno essere applicate in maniera più snella, più efficace e rispondente agli scopi e al dettato della disciplina dell'articolo 3.

un numero sostanzioso di palazzi di impostazione rinascimentale, ricostruiti ai primi del Settecento, dopo il terremoto del 1703,

quindi un impegno, dopo il primo passo fatto in Commissione, a mettere al centro delle preoccupazioni questa enorme questione. si reca all'Aquila in questi giorni, vedrà che la città fa ancora impressione malgrado i lavori di primo intervento: non c'è nessuno. Questo è un punto centrale per la ricostruzione.

costituisce una modifica al testo originario approvata in Commissione dopo ampio dibattito e con il consenso di quasi tutte le forze politiche presenti.

Quindi le abitazioni principali vengono interamente risarcite del danno che hanno subito. Questo è un momento importante, come si è sottolineato in più interventi, perché si accerta con chiarezza questo punto. L'altro punto di chiarezza che è scaturito dalla discussione riguarda l'utilizzo del credito d'imposta, che avviene su richiesta dell'interessato, quindi la discrezionalità è riservata al beneficiario e, per un'ulteriore interpretazione, ritengo di poter affermare che il credito d'imposta, sempre su base volontaria, sia utilizzabile anche in occasione di eventuale ammortamento di finanziamenti agevolati.

intervenire ulteriormente in favore di quei cittadini che, nella normalità della loro attività e della loro sistemazione familiare, avevano deciso di acquistare un'abitazione principale; lo avevano fatto fatto accendendo un mutuo e quindi sicuramente avevano e hanno un debito residuo. Lo Stato interviene su questo debito residuo

del Governo sia in termini di chiarezza, rispetto ai contributi e all'utilizzo del credito d'imposta, sia in termini di risorse, perché sicuramente saranno moltissimi i cittadini e i nuclei familiari che beneficeranno di questa ulteriore previsione.

su cui ho espresso parere contrario intervengono su aspetti della ripresa economica (l'attivazione di imprese e così elaborare un ordine del giorno che non mancherà di trovare non solo l'approvazione del relatore e del Governo, ma, credo, anche la condivisione di tutte le forze politiche. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno

3.717 sarebbe forse più opportuno un ordine del giorno, che sarebbe sicuramente condiviso da tutte le forze politiche: infatti, questi emendamenti, a partire da questo presentato dal senatore Lusi, per seguire con i successivi, affrontano il problema sicuramente importante e sensibile delle condizioni di disagio economico in cui si vengono a trovare le aziende municipalizzate e gli stessi comuni. Come ho detto, siamo ancora in una fase di emergenza per cui non è quantificabile questo tipo di disagio e quindi sarebbe più opportuno che il Senato impegnasse il Governo a riferire sull'argomento e a prendere importanti decisioni in merito quando si avrà un quadro completo del disagio economico che comuni e società municipalizzate hanno subito a seguito del terremoto. Non vi è dubbio che, così come assistiamo i cittadini, i proprietari dell'abitazione principale e i beni storico-culturali e così come andremo ad assistere le imprese, dobbiamo anche assistere quelle imprese che, essendo pubbliche, forniscono soprattutto servizi. credo sia prematuro affrontare oggi il discorso e quindi ritengo che, anche su questo argomento, che è stato sollevato ed è importante, si possa convenire sulla stesura e l'approvazione di un ordine del giorno che sia impegnativo per il Governo per esaminare, come ho già detto, interventi a favore dei comuni e delle aziende municipalizzate non appena il quadro sarà chiaro.

3.321, anche perché entra nel merito della modalità di corresponsione dei contributi e questo sarebbe meglio fosse riservato alle ordinanze. Ho più volte cercato di inquadrare il contesto normativo in cui si muove questo decreto, sottolineando che esso dà le linee guida e gli indirizzi, stabilisce alcuni limiti e tipologie e poi le ordinanze passano alla fase applicativa. L'argomento dell'emendamento

che sono emesse con il concerto del Ministero dell'economia, disciplineranno l'utilizzo dell'eventuale quota di credito d'imposta non immediatamente assorbita a copertura del contributo.

3.328 mi sembra assolutamente ultroneo, anzi, direi quasi fuori dalle previsioni adottate e quindi il parere è contrario. Il parere è contrario volendo, in un ordine del giorno, ma rientra in quel ragionamento che facevo poco fa, in ordine alla gestione delle società municipalizzate.

tecnicamente proponibile. Vi è anche, peraltro, un subemendamento del relatore all'emendamento approvato in Commissione, che propone la corresponsione delle sovvenzioni per la zona franca in ambito triennale, non solamente per il 2009 come approvato in Commissione, ma anche per il 2010

3.700 per affrontare un problema che in realtà l'Aula ha già sfiorato quando è stato proposto l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 3.

definisce - sarebbe meglio dire definiva, perché ormai il lavoro molto positivo della Commissione ha modificato queste provvidenze a favore dei terremotati - un intervento a favore delle attività di ricostruzione delle abitazioni e degli opifici interamente distrutti o gravissimamente danneggiati e in ogni caso inagibili. Quell'intervento viene finanziato con una serie di misure di aumento delle entrate (con particolare riferimento alle entrate da prelievo fiscale sui giochi) poi coperto fondamentalmente facendo riferimento alle risorse contenute nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e di cui noi abbiamo avuto conto, da parte del Governo, con relazione tecnica regolarmente asseverata dal Ragioniere, che oggi dispone di una cifra molto ingente e pienamente disponibile (cioè non impegnata) di circa 7 miliardi di euro. Le provvidenze disposte in particolare dall'articolo 3 del decreto-legge originario venivano dunque coperte con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, che si riferisce, appunto, all'uso delle risorse del Fondo strategico per il Paese.

modifica in modo integrale, estendendoli, gli interventi a favore della ricostruzione delle case prima abitazione e degli opifici, stabilendo esplicitamente la concessione di contributi a fondo perduto,

del testo del decreto originariamente emanato dal Consiglio dei ministri, con la quale si assicurano due cose: anzitutto, che il contributo è a fondo perduto luogo, che quel contributo a fondo perduto copre interamente l'onere della ricostruzione. È del tutto evidente - del resto, se fosse diversamente, non si capirebbe perché la Commissione abbia approvato quell'emendamento - che questa norma modifica

a quel Fondo si attingeva da 2 a 4 miliardi con le vecchie provvidenze (certamente inferiori rispetto a quelle disposte dall'emendamento approvato in Commissione),

Siccome il Governo ha riferito in Commissione bilancio che su quel fondo non ci sono soltanto 4 miliardi di euro, ma ce ne sono 7 non non impegnati (quindi disponibili), è del tutto evidente, signor Presidente, che la proposta di discutere tutti questi emendamenti soltanto dopo che la Commissione bilancio abbia espresso il suo parere sull'emendamento della Commissione che quel che vale per l'emendamento della Commissione vale per tutti gli altri. Se sono disponibili fino a 7 miliardi è ovvio che se le provvidenze aumentano bisognerà che nell'articolo 14, comma 1, il riferimento sia da, almeno, 3 miliardi di euro a 5, 6, 7 miliardi in rapporto alla valutazione circa l'entità dei costi da sopportare per aumentare le provvidenze da X, così come erano disposte nel testo originario del decreto, a X più Y, così come sono disposte ora dal testo licenziato dalla Commissione. Questo è il punto che avrebbe suggerito, come misura di buon senso, di discutere di tutti gli emendamenti all'articolo 3, compreso quello della Commissione, soltanto dopo che il Governo avesse accettato

momento le stesse risorse sono assegnabili a due finalità completamente diverse. Ma è del tutto evidente che una delle due finalità non sarebbe perseguibile. Questo a me sembra soltanto un ragionamento di buon senso quindi è palese che se vogliamo affrontare in termini di ordine logico l'argomento al nostro esame, dobbiamo conoscere il parere della Commissione bilancio sulla base della relazione tecnica sull'emendamento della Commissione che poi finirebbe per riguardare interi emendamenti, perché tutti si coprono sul comma 1 dell'articolo 14, come è inesorabile. Signor Presidente, termino con un'osservazione. Se si dice «fondo perduto» per coprire l'integrale costo dell'intervento, lei mi sa dire per quale ragione una persona che si comporti razionalmente dovrebbe far riferimento al credito d'imposta sulle imposte che dovrà pagare da qui al 2032? L'economia, come lei sa, sbagliando presuppone comportamenti razionali e questo è certamente sbagliato ed è la ragione per la quale gli economisti sono noti per essere quelli che dopo dieci anni spiegano perché dieci anni prima si erano sbagliati, come disse il maestro di tutti gli economisti.

Io penso che per quanto si possa dar spazio al comportamento irrazionale, non ci sarà nessun cittadino dell'Abruzzo colpito dal terremoto che ricorrerà a questa misura. Il che vuol dire, signor Presidente, che nel 2009‑2010 dovremo avere a disposizione tutte le risorse necessarie. Ma questo solleva un problema di grande portata. Quel Fondo è un fondo strategico costituito per interventi le cui risorse - apprendiamo - a metà 2009

Ma allora, in termini di cassa, signor Presidente, nel 2009 e nel 2010 di quei 7 miliardi che sono disponibili nel Fondo se a metà del 2009 non abbiamo neanche programmato cosa farne, quanti ne avremmo spesi se non ci fosse stato il terremoto d'Abruzzo e non avessimo impiegato quelle risorse per l'intervento a favore delle provvidenze sul terremoto? Ne avremmo speso una quota molto limitata perché lei sa che c'è un coefficiente di realizzazione della spesa in conto capitale

della sostanza del provvedimento al nostro esame si pongono due problemi. Innanzi tutto, se non c'è la relazione tecnica sul nuovo emendamento approvato dalla Commissione è evidente che stiamo discutendo completamente al buio, in un contesto nel quale potremmo stare impegnati ad approvare una norma che già oggi non ha più la copertura necessaria, copertura che si può e si deve trovare alzando quei 4 miliardi fino a 5, 6, o quanto necessario: tanto ce ne sono 7, e certamente possiamo utilizzare luogo, per un problema di trasparenza, non è serio di fronte al Paese che a metà del 2009 si dica che nel bilancio dello Stato ci sono 7 miliardi di euro impiegabili immediatamente che oggi non sono destinati a fare nulla, perché se non sono destinati a fare nulla l'argomento che ho usato a proposito del rapporto tra competenza giuridica e cassa viene accentuato ed esasperato in modo assolutamente intollerabile. non sono destinate a far nulla vuol dire che non si sarebbero spese, ma se non si fossero spese noi, impiegandoli per un intervento immediato sul terremoto, stiamo facendo un'operazione che dal punto di vista della cassa è completamente scoperta.

Il collega Morando pone nel merito due problemi sui quali si è discusso con grande profondità e che la Commissione da me presieduta ha ritenuto così significativi da dover richiedere una relazione tecnica al Governo, in particolare sulla prima delle due questioni poste, che provo a riassumere. C'erano delle provvidenze per le quali il Governo stimava una cifra da 2 a 4 miliardi di euro;

Tale questione è stata ritenuta così rilevante all'interno della Commissione che abbiamo chiesto la relazione tecnica al Governo esattamente su quel punto, perché non vi è dubbio onestamente che la misura delle provvidenze comporta necessariamente un tetto più elevato. La seconda questione è ancora di critica ad una risposta puntuale del Governo in Commissione, ovvero che su quel Fondo

Sul piano del merito ribadisco che il Governo in Aula ha detto che non sono impegnati e quindi vale la prima delle due considerazioni: se non sono impegnati, e dunque ci sono 7,5 miliardi, una quota degli stessi può essere usata per aumentare il tetto massimo di quelle provvidenze che con questo emendamento vengono aumentate. Mi sembra di aver riassunto con puntualità le critiche del senatore Morando.

punto, le questioni sulla copertura saranno integralmente affrontate in quella sede nella quale, poiché in quest'Aula non si vota l'articolo, certamente verrà modificato l'impianto dell'articolo ove il Governo acceda alla richiesta fatta dai senatori. Solo per questo, signor Presidente, insisto per la questione di metodo, affermando che è possibile procedere perché questi significativi problemi

**Il Senato non approva.**

**Il Senato non approva.**

vengono respinti semplicemente perché è ovvio che le attività produttive di beni e servizi sono tutte comprese? Credo che una precisazione del genere sia rilevante ai fini dell'interpretazione sul contenuto della norma.

non entrano più le risorse per far fronte al pagamento degli stipendi. Il Comune dell'Aquila e i vari Comuni del cratere avranno perdite,

affrontare un provvedimento di questo tipo senza porsi il problema dei comuni e della province, insomma degli enti locali in genere, e delle società pubbliche, che rischiano il dissesto finanziario?

sono della stessa opinione del relatore. Voglio rimarcare, esprimendo un concetto più generale, che tanto il Governo quanto il relatore sono stati molto attenti

della nostra posizione politica. Domani mattina i sindaci di quei Comuni e i presidenti di quelle aziende non sapranno come pagare gli stipendi ai lavoratori!

se non lo volete affrontare, presentatelo voi un ordine del giorno. Noi vogliamo votare e voi vi assumerete le vostre responsabilità nei confronti di tutti i dipendenti di quegli enti locali, dei fornitori, dei sindaci e di tutti quanti hanno la responsabilità di erogare servizi pubblici, tutti i giorni, senza soldi.

Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento e credo che sia opportuna una riflessione in questo senso, perché quando si vuole le risorse si trovano. Ricordo a me stesso che questa maggioranza e questo Parlamento hanno trovato risorse per 500 milioni di euro in favore del Comune di Roma,

80 milioni di euro. Io credo che la situazione eccezionale nella quale si trovano i Comuni interessati dal terremoto, e in particolar modo il Comune capoluogo, meriti un'attenzione e una sensibilità, se si mi è consentito, maggiore proprio in questo momento.

tacciati di usare lo «spannometro», quale può essere un primo intervento utile, anche sulla base degli esiti del dibattito sull'articolo 14, laddove si chiariranno esattamente i contenuti anche economici complessivi e finanziari dell'intero provvedimento, figuratevi se sarò io ad

è un'altra cosa

Noi partiamo dall'assunto - ne discuteremo e le ragioni sono state ampiamente illustrate dal collega Morando - dell'insufficienza delle risorse per

grave carenza di risorse finanziarie. Sosteniamo cioè che almeno, se non si integra la risorsa complessiva nei termini che abbiamo chiesto, per il 2009 dobbiamo anticipare una quota a richiesta, pari al 30 per cento, per avviare la ricostruzione. C'entra eccome con il cuore del problema, cioè la sufficienza o no delle risorse per avviare la ricostruzione! Quindi, stiamo chiedendo un accantonamento perché, se troviamo un'intesa sulla prima parte, ritireremo questi emendamenti; altrimenti, chiederemo che essi vengano votati.

per dire al collega Legnini che è impossibile sostituire le anticipazioni di cassa del bilancio dello Stato con anticipazioni soggettive rispetto ai possibili beneficiari. Ritengo che ci siano gli elementi perché già nel 2009 si possano avere le risorse per finanziare la capacità di spesa che saremo capaci di mettere in campo e credo che questa sia una cosa sacrosanta. La metodologia

un mondo di problemi rispetto ai beneficiari. Credo che sia opportuno concludere l'*iter* perché, comunque, ci saranno risorse nel 2009 - è stato ampiamente assicurato - e tutti potranno ricostruire la loro casa o fare gli interventi di cui possono beneficiare presentando le fatture in banca e ottenendo, di conseguenza, immediatamente l'erogazione.

i loro comportamenti; lo abbiamo denunciato ieri: alcune banche hanno addirittura revocato le carte di credito perché non si fidano dei terremotati. Questo emendamento

come questo, che è di interesse generale, anche perché, lo ripeto, queste banche - ieri lo ha detto anche il Ministero dell'economia - dovrebbero abbassare i tassi; fanno la cresta sui conti, hanno le condizioni più onerose ed i costi dei conti correnti più alti d'Europa: perdono il pelo ma non il vizio. È un emendamento di buonsenso. Quindi, chiedo

delle somme stanziate per la ricostruzione andranno ai professionisti. Vogliamo applicare le tariffe massime anche se i progetti spesso vengono ripetuti da un paese all'altro? Non sarebbe opportuno delegare il commissario a dimezzare le tariffe relative

approfondire la questione in quanto può essere possibile riformulare meglio questo emendamento, che non ha costi per le pubbliche amministrazioni e per lo Stato e consente nella ricostruzione, qualora ci sia l'accordo dell'amministrazione comunale, il trasferimento di cubatura laddove si individui magari nella vecchia composizione del tessuto urbano una opportunità di creare spazio a servizi, a verde o a parcheggi che siano di pubblico interesse e che quindi siano realizzabili spostando la volumetria.

Signor Presidente, prendo la parola per comunicare che nei giorni scorsi Taiwan è stata invitata a partecipare in qualità di osservatore all'Assemblea mondiale della sanità che si è aperta il 18 maggio scorso a Ginevra. Questo traguardo è stato raggiunto dopo ben 12 anni di sforzi e una solidarietà che ha visto partecipi tanti liberi Parlamenti, tra i quali il nostro - voglio sottolinearlo - quello europeo e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, che recentemente ha votato all'unanimità una mozione pro Taiwan. un traguardo nell'interesse della salute dei diritti umani, non soltanto dei 23 milioni di cittadini taiwanesi, bensì di tutta l'umanità. È stato possibile arrivare a tale importante risultato grazie alla pragmatica politica di dialogo e di collaborazione avviata dai Governi di Taipei e Pechino, della quale si aveva parlato il presidente del Parlamento di Taiwan, onorevole Wang, nella sua visita al nostro presidente Schifani lo scorso 3 febbraio. Una nuova politica da incoraggiare e sostenere, che in pochi mesi ha rotto il muro attraverso lo stretto di Taiwan e che oggi vede l'isola collegata al continente da ben 270 voli settimanali. Auspico che la soluzione adottata in seno all'Assemblea mondiale della sanità con la denominazione *Chinese Taipei*, già da anni in vigore nel Comitato olimpico internazionale e nella Conferenza economica dell'Asia-Pacifico, sia presto adottata anche in tutti gli altri fori multilaterali internazionali - penso ad esempio alla FAO che opera da Roma - nei quali Taiwan può e deve dare il suo significativo contributo al bene comune. Per questi motivi, signor Presidente annuncio il ritiro della mozione che avevo promosso per impegnare il nostro Governo a sostenere la partecipazione come osservatore di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità. Ringrazio i colleghi senatori, anzitutto il presidente Gasparri, che avevano condiviso e sostenuto questa giusta finalità. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fatto personale alla fine della seduta, come previsto peraltro dal Regolamento, anche per non perdere ulteriore tempo durante i lavori dell'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto. Signor Presidente, il sottosegretario Menia, presente in rappresentanza del Governo, si è permesso di usare una frase nei confronti dei parlamentari, in particolare di coloro che stavano illustrando gli emendamenti, che non è concessa a nessun membro del Governo.

quando si riferiva alla parola nullo, si rivolgeva ad un comportamento politicamente nullo del Sottosegretario che rappresenta il Governo. Egli rappresenta il Governo di questo Paese, non rappresenta se stesso. Signor Presidente, questo andava censurato, ancorché nelle forme lievi e sempre politicamente parlando, perché nessun rappresentante del Governo può dire Governo può dire ad un parlamentare che nell'esercizio del suo mandato sta esagerando o sta andando fuori misura, a meno che questo non sia vero e, nella fattispecie, non lo era.